Presidente, onorevoli senatrici e senatori, il presente disegno di legge è composto da cinque articoli ed è stato esaminato in sede referente dalla 7a Commissione dal 28 gennaio 2014 al 30 settembre 2015. In sintesi, l'obiettivo che si propone è di uniformare la disciplina dei limiti al rinnovo dei mandati degli organi di vertice del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato paralimpico (CIP), delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva. Annuncio, in sede di presentazione dei contenuti del disegno di legge, il deposito di alcuni emendamenti volti a sostituire l'attuale formulazione degli articoli 1 e 2. In particolare, l'emendamento proposto all'articolo 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 242 del 1999. La disposizione consente agli organi del CONI di restare in carica quattro anni e i componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e alcuni componenti della giunta nazionale, ovvero 10 rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, il rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva e i due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI non possono svolgere oltre tre mandati. Si propone, inoltre, l'estensione di tale disciplina anche al presidente e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI. In base all'articolo 4, comma 1, il CONI adegua il proprio statuto alle disposizioni appena richiamate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, l'autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i quindici giorni successivi, dichiara decaduti i componenti degli organi del CONI sprovvisti dei requisiti di legge per la permanenza in carica. Una disciplina di tenore sostanzialmente analogo viene introdotta dall'emendamento proposto all'articolo 2, che modifica il comma 2 dell'articolo 16

La disposizione assegna agli statuti il compito di prevedere le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, i quali restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati. La norma vigente, che si intende abrogare (l'abrogazione esplicita è prevista all'articolo 5, comma 2, del presente disegno di legge), prevede la possibilità della riconferma per la carica di presidente, sancendo la non immediata rieleggibilità alla suddetta carica per chi abbia ricoperto due mandati consecutivi, salvo che non si raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti validamente espressi. In tal caso non vi sono limiti alla possibilità di riconferma. La disciplina proposta con la modifica della suddetta norma stabilisce invece che, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee federali, entro quattro mesi dalla data di entrata in in vigore della presente legge, il CONI stabilisca, con proprio provvedimento, i criteri di esercizio del diritto di voto per delega in assemblea per limitare la concentrazione delle deleghe, mediante una revisione del massimo di quelle che possono essere rilasciate e che non supera, in ogni caso, il numero di Vale la pena richiamare la deliberazione del consiglio nazionale del CONI n. 1523 del 28 ottobre 2014 che prevede, attualmente, nell'ambito dei principi assembleari, un numero massimo di deleghe tra società e associazioni sportive pari a 40. La stessa deliberazione, che contiene i principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, prevede, per quanto concerne l'assemblea ordinaria elettiva, che entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi debbano essere svolte le assemblee ordinarie elettive da parte delle federazioni Quelle che, invece, partecipano ai giochi invernali provvedono alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea entro tre mesi dalla chiusura dei giochi. Aperta questa breve parentesi esplicativa e ritornando alla disciplina proposta nel disegno di legge si stabilisce che, a fronte di un eventuale inadempimento federale alle disposizioni del CONI da adottare entro quattro mesi dalla data di approvazione del provvedimento *ad hoc* del CONI, quest'ultimo ente nomini un commissario *ad acta* che provvede entro sessanta giorni alla nomina. Resta ferma la possibilità per gli statuti federali di prevedere un numero di mandati inferiore al limite stabilito dal nuovo comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. È previsto, infine, che la disciplina appena illustrata si applichi anche agli enti di promozione sportiva e al presidente e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. L'articolo 2-*bis* del disegno di legge, che modifica l'articolo 3 della legge n. 189 del 2003 aggiungendo l'articolo 3-*bis*, estende la normativa contenuta negli articoli 1 e 2 del presente progetto di legge al Comitato italiano paralimpico e alle federazioni sportive nazionali paralimpiche e discipline sportive associate. Infine, l'articolo 4 del disegno di legge, comma 4, in materia di disposizioni transitorie, prevede che tutti coloro che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, se eletti, possano svolgere ulteriori due mandati. L'articolo 5, comma 1, abroga

al numero dei mandati possibili al presidente e ai membri degli organi territoriali del CONI, al presidente e ai membri degli organi direttivi, nazionali e territoriali, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, nonché agli enti di promozione sportiva; nella sostanza, a tutta la *governance* sportiva, le cui regole fino ad ora hanno permesso - è il caso di molti presidenti federali - una permanenza in carica oltre modo lunga. La percentuale minima del 55 per cento, infatti, prevista dalla legge dal terzo mandato in poi, non ha rappresentato, di fatto, un ostacolo un ostacolo alle rielezioni multiple, comportando il rischio che le risorse federali fossero investite per la rielezione degli organi di vertice piuttosto che per il raggiungimento di obiettivi tecnici e per la promozione dello sport. Compito delle federazioni, invece, invece, è promuovere e sviluppare la preparazione psico-fisica degli atleti nelle singole discipline sportive a carattere agonistico e amatoriale, in armonia con gli indirizzi del CIO e del CONI, curando la preparazione tecnica, didattica e metodologica dei tecnici sportivi e realizzando e organizzando attività sportive specifiche, sia di avviamento allo sport sia di sport di alto livello. Conviene concludere con alcune brevi considerazioni. L'estensione del limite di tre mandati per presidente e componenti della giunta nazionale del CONI è in linea con la durata in carica del presidente del il Comitato olimpico internazionale. La carta olimpica prevede, difatti, la permanenza in carica del presidente per otto anni, rinnovabili una sola volta per quattro. In questo modo l'ordinamento nazionale si adegua a quello sportivo internazionale, permettendo agli organi di vertice del CONI e delle federazioni di costruire i rapporti a livello internazionale e di incidere su tali politiche. Aspetto, poi, senz'altro rilevante è quello di garantire un *turnover* finora bloccato all'interno delle federazioni sportive nazionali, dove ci sono presidenti in carica dagli anni Novanta o dagli inizi del nuovo millennio, che - in alcuni casi eclatanti giunti alla ribalta delle cronache nazionali - hanno beneficiato di veri e propri stratagemmi elettorali utili per la loro rielezione e legati alla creazione e alla gestione di associazioni e società sportive affiliate alle federazioni, in realtà fasulle, utilizzate come bacino di voti in occasione delle assemblee elettive federali, tramite il voto per delega. Di casi, purtroppo, ve ne sono stati parecchi. Quello che ha coinvolto i vertici della federazione del pentathlon in tempi recenti è uno dei più noti. Infine, ricordo la necessità di una disciplina transitoria nei termini proposti, assolutamente necessaria al fine di evitare che le nuove disposizioni possano contravvenire al principio generale sancito dall'articolo 11, primo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile che, in materia di efficacia della legge nel tempo, dispone che essa non possa avere effetto retroattivo. Per tale ragione, si stabilisce che i limiti previsti dalla nuova normativa non si applichino a chi è in carica alla data di entrata in vigore della legge che, se eletto, può svolgere altri due mandati. Questo significa che tutti partiranno da zero, potendo svolgere tre mandati, ma chi è già in carica non può svolgerne più di altri due, partendo dal presupposto che, dei tre consentiti dalla nuova normativa, almeno uno sia già in corso. In sostanza, appena entra in vigore la legge - ed è indispensabile che lo sia in tempi brevissimi - si riparte tutti, vecchi e nuovi, da zero, ma questa volta con limiti certi, definiti e non derogabili. Fatta salva la normativa transitoria si stabilisce, quindi, che, nel tempo massimo di otto anni, si sarà verificato un ricambio totale dell'attuale *governance* politica del mondo sportivo e, attraverso i tre mandati, si garantisce allo sport italiano una presenza efficace nella politica sportiva internazionale.

Signora Presidente, il presente disegno di legge giunge opportunamente a ripristinare i limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano e delle altre federazioni sportive nazionali, già previsti dalla disciplina originaria del decreto legislativo n. 242 del 1999, il quale prevedeva che non potessero essere esercitati più di due mandati. Nel 2004 - com'è noto - è intervenuta una disciplina transitoria che, fino ad oggi, ha permesso il rinnovo continuo dei mandati ben oltre gli otto anni, anche al di fuori dei casi specificamente previsti dalla normativa. Tale situazione ha reso necessario l'intervento legislativo in oggetto, al fine di ristabilire una disciplina più equa e rispondente al mutato quadro legislativo ed economico-sociale nazionale e internazionale. È da rilevare, inoltre, che il testo approvato dalla 7a Commissione è stato significativamente modificato rispetto al disegno di legge originario, a seguito di un interessante *iter* di consultazione degli organi interessati, che si è svolto nell'arco di circa un anno. Gli aspetti più significativi riguardano l'applicazione delle limitazioni

i lavori della Commissione hanno evidenziato alcune criticità, soprattutto relative alle federazioni molto piccole, per le quali talvolta risulta difficile trovare dei successori negli organi direttivi. Tuttavia, nonostante gli approfondimenti svolti con le strutture territoriali delle diverse società interessate, non è stato ritenuto opportuno introdurre diversificazioni, anche perché in alcuni casi la presunta impossibilità di trovare candidati può essere utilizzata come strumento per rimandare innovazioni legislative. Lo sport, quindi, come pratica di massa, costume sociale e utilità finalizzata all'implementazione del tasso di salute nella popolazione, è destinato ad avere sempre più rilevanza nel mondo e, in particolare, nel nostro Paese. Fenomeno complesso, di grande impatto sull'economia, sulla società, sui sistemi del volontariato, sul terzo settore, sull'imprenditoria e sui programmi della pubblica amministrazione, la pratica sportiva richiede sempre più capacità di *governance*, gestione oculata e manageriale mediazione permanente tra esigenze di democrazia partecipata e finalizzazione all'ottimizzazione dei risultati fisici e morali degli atleti.

degli obiettivi richiederà sempre più presenza attiva e operativa sui tavoli decisori, sui campi, sulle piste e sugli impianti di gara. Lo sport italiano deve ancora superare il *gap* atavico tra Nord e Sud del Paese, tra Centro-Nord e Centro-Sud, con la parte settentrionale dell'Italia in minore sofferenza rispetto alle situazioni, talvolta arcaiche, in cui nel Mezzogiorno, meno favorito e sostenuto dai sistemi sociali ed economici, la pratica sportiva si svolge con difficoltà. Sarebbero opportune fasi di approccio culturale intermedio, preparatorie delle nuove sfide, e dei nuovi bisogni e tendenze sociali:

Pertanto, la dirigenza, a tutti i livelli applicata, oltre che appassionata deve accompagnarsi a competenze, inclinazioni all'ascolto e predisposizione alla partecipazione. Nei mandati che il Parlamento si accinge a statuire per i Presidenti di federazione, questi requisiti devono essere rispettati. Nella lunga stagione della candidatura a ospitare a Roma le Olimpiadi del 2024 sarebbe auspicabile che le federazioni sportive e il CONI mostrassero al Paese consapevolezza del proprio ruolo e tendenza ad accogliere il vento nuovo che spira nelle periferie e sui campi sportivi.

retroattivi oppure no. Un serio dibattito sullo sport italiano richiede altro. Provo a spiegarmi. Ritengo importante che un'Assemblea come la nostra Il CONI nasce in Italia nel 1908, come associazione dei rappresentanti dei vari sport, al fine di preparare ed assistere la partecipazione italiana alle olimpiadi. Nel 1927 si decide l'accorpamento di tutte le federazioni sportive e infine, con la legge n. 426 del 6 febbraio 1942, il CONI viene riconosciuto dallo Stato come ente dotato di personalità giuridica, preposto alla cura, all'organizzazione e allo sviluppo dello sport.

È un ente pubblico non economico, posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, con delega all'erogazione di contributi statali alle federazioni sportive nazionali e a quelle associate, che non possono accedere direttamente ai finanziamenti perché enti di diritto privato. Ritengo che nella vita di tali organismi attualmente lo Stato eserciti un ruolo molto indiretto e per questo trovo poco corretto, anzi lesivo dell'autonomia degli enti stessi, che sia lo Stato a dover decidere il numero dei mandati degli organi direttivi. Per giunta questo non accade in alcun altro Paese europeo comparabile con l'Italia. Anzi, all'estero spesso è lo Stato che eroga direttamente i contributi alle federazioni. La questione non è secondaria. Perché in Italia, un Paese che si è sempre distinto in ogni competizione, ad ogni livello e in tutte le discipline, l'organizzazione del progetto sport non è affidata ad un Ministero *ad hoc*, che si occupi della pratica sportiva, del suo sviluppo e della capillare diffusione della cultura sportiva? Non vi è chi non colga la disparità di valorizzazione che c'è attualmente tra ogni ente locale, che si dota di assessorati allo sport e simili, e uno Stato sovrano che non dedica un Dicastero ad uno degli *asset* più prosperi, più seguiti, più aggreganti più aggreganti (e potrei trovare altre decine di aggettivi) della nostra società. Si era tornati a parlare di un Ministero per lo sport qualche anno fa, magari naturale destinatario del famoso tesoretto derivante dagli incassi il CONI avrebbe dovuto solo occuparsi dell'attività olimpica, cioè della partecipazione e dell'immagine del nostro Paese al più grande evento sportivo planetario, non anche della direzione e della visione che un Paese vuol dare ai cittadini in una materia tanto importante e di cui ci ricordiamo solo - e spesso, per fortuna - quando i nostri campioni si distinguono in tutto il mondo. dimentica, in tali occasioni, che esiste una rete territoriale fatta di giovani che hanno difficoltà ad avere accesso alle pratiche sportive, se non innanzitutto al primo avviamento alla pratica sportiva. Esiste uno sport giovanile trascurato e abbandonato ed esiste lo sport di base, che è completamente sostenuto dalle famiglie, indipendentemente dal loro censo; lo sport sociale, la redistribuzione territoriale di strutture e risorse economiche, la prevenzione, l'impiantistica, la scuola. Non spetta forse allo Stato una simile organizzazione o, almeno, indicarne le linee programmatiche e di sviluppo? Vedete, colleghi, questo tema mi sta particolarmente a cuore. Dunque per me il problema sui limiti dei mandati degli organi del CONI non è il centro della questione. Le vere difficoltà dipendono dalla sua particolare natura e collocazione Un esempio per tutti: il CONI dal 2002 si avvale della collaborazione della CONI Servizi SpA, mediante un contratto annuale nel quale vengono identificati gli obiettivi e i risultati da raggiungere. Fra i compiti della CONI Servizi SpA, c'è anche quello di risanare i bilanci del Comitato olimpico nazionale. Piuttosto, siccome di quattrini pubblici si tratta, non sarebbe più interessante conoscere gli esiti dei controlli eseguiti da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato dei servizi ispettivi - nei confronti del CONI e delle sue federazioni in merito alla gestione finanziaria di queste ultime? Non sarà piuttosto interessante scoprire chi lavora bene e chi invece crea debito alla propria federazione? Eventualmente, di quest'ultimo dovrebbe essere sancita per legge l'automatica decadenza, Osservo che gli estensori di questa nuova norma che ci apprestiamo a votare hanno fatto riferimento, *excusatio non petita*, ad una formula che già considera intoccabile lo *status quo*. Leggo infatti: «Fermo restando il rispetto per l'autonomia gestionale del CONI». No, onorevoli colleghi, si tratta, come ripeto, di quattrini pubblici, non di autonomia gestionale delle risorse, ed anche di pubblico interesse. Confermo che nella legge si pone una questione di cristallizzazioni nell'assetto gestionale. Ma in un frangente politico ed economico come quello attuale, possiamo sorvolare sulla effettiva funzionalità di un ente nato nel 1908 per preparare le Olimpiadi e che da più parti viene considerato come superato, se non addirittura discusso e anarchicamente condotto da più di un secolo? Possiamo sottrarci all'esercizio della nostra responsabilità di legislatori? Possiamo avallare ancora una situazione ben lontana dall'essere trasparente e virtuosa, limitando la discussione al numero dei mandati? Quanti dei cospicui fondi che il CONI, come ente pubblico, riceve dallo Stato e che poi distribuisce alle federazioni vengono veramente impiegati per l'attività sportiva? E quanti invece vengono spesi in burocrazia e politica dello sport? Magari sarà il caso di riprendere in mano quello studio del professor Roberto Perotti, peraltro commissionato tempo addietro proprio dal *premier* Renzi, sui *manager* degli enti pubblici, che definiva CONI Servizi, ironicamente,

«Un modo semplice ma non molto sottile» asseriva Perotti «per creare stipendi». Insomma, secondo l'illustre tecnico, autore di una relazione mai smentita (poi dimessosi perché forse non aveva ottenuto effetti), si tratta di un vero e proprio pozzo senza fondo per stipendi, incarichi, consulenze e poltrone.

con un presidente e un amministratore delegato che decidono le sorti e le finanze del nostro sport assieme ad un numero di consulenti incredibile, tra avvocati, direttori di lavori, medici per i referti, docenti per i corsi? Simili enti non li avremmo forse definiti carrozzoni, ai tempi in cui la «casta» sembrava abitare solo quest'Aula? Per carità, Dio salvi le Olimpiadi. Anche se mi dicono che nessuno ha ancora visto uno straccio di bilancio sul precedente comitato olimpico, quello per Roma 2020. E chi di noi, poi, non ha gioito per la memorabile *performance* qualche giorno fa della nostra nazionale di calcio? Vi sarà chiaro che la sportività non entra in queste mie puntualizzazioni. E mi mi rifiuto di pensare che possiamo continuare ad assistere ad un intensivo utilizzo di danari destinati anche alle attività sportive minori per mandare avanti una costosa ed elefantiaca macchina che di soldi ne dovrebbe produrre, invece, per destinarli magari allo sviluppo della pratica e della cultura dello sport e del benessere, prima ancora che all'attività sportiva puramente agonistica. Nel 2012, anno analizzato dalla Corte dei conti, durante il quale sono emersi irregolarità e sprechi rilevanti, il CONI disponeva di risorse per 428 milioni di euro (di cui 408,9 provenienti dal Ministero dell'economia e e ha versato a federazioni, discipline associate, enti di promozione sportiva e Forze armate circa 246 milioni. Il resto, cioè la bella cifra di 182 milioni di euro, serve infatti al funzionamento del CONI stesso.

milioni) sono destinati al «progetto di alfabetizzazione motoria» nelle scuole primarie, varato insieme al MIUR. Un investimento che non può certo considerarsi sufficiente a diffondere una vera cultura sportiva in famiglia, a scuola, nella società. Una società in cui un bambino possa sviluppare le proprie abilità motorie - tutte - per poi specializzarsi, eventualmente, in una disciplina. Ma sembra quasi che al CONI e alle federazioni e ai loro dirigenti, alcuni dei quali restano lì decenni e decenni, questo non interessi. Così oggi nella civilissima Italia, ai primi posti per progresso e cultura, solo la metà dei bambini pratica sport (due volte a settimana) e il 23 per cento tra i sei e gli undici anni ha problemi di obesità. A conti fatti, restano, tanto per precisione e per chiudere il discorso, oltre 130 milioni di euro che - quelli sì - mi piacerebbe vedere documentati. Il mondo dello sport è certamente un *asset i*mprescindibile. Al centro di questo mondo ci dovrebbero essere tutti gli individui, di ogni età, genere, estrazione sociale, capacità motoria e intellettiva; lo sport per tutti, in virtù degli aspetti salutistici dell'attività motoria, intesa come fattore di prevenzione, miglioramento della qualità della vita e riduzione della spesa pubblica. È necessario vedere pienamente coinvolti tutti i soggetti competenti in materia, in una virtuosa sussidiarietà sociale. Potremmo essere un Paese esempio per gli altri d'Europa, sia per la qualità dei nostri sportivi, sia per le caratteristiche della struttura geografica del nostro Paese, che per clima, storia, paesaggi e cultura, non ci limita in alcunché. Sono condizioni uniche al mondo. Colleghi, noi invece siamo fermi al CONI, alle federazioni, alle cariche sociali, alle bizzarre e cervellotiche modalità elettorali (il 55 per cento al terzo mandato, altre percentuali per altri mandati), agli spazi da creare per trombati eccellenti e, infine, al numero dei mandati. A proposito, questi mandati verranno svolti a titolo gratuito e senza conflitto di interessi, come solennemente dichiarano tutti gli statuti federali? O saranno documentati in altro modo, magari mascherati da incarichi e consulenze in CONI Servizi? Ci sarà una ragione, ed è una ragione che sarà difficile da spiegare a quei nostri giovani concittadini che, allenandosi con con un canestro artigianale o lanciando una pallina al di là di una rete, avrebbero potuto diventare cittadini migliori e, forse, i campioni che domani potremmo non avere più. Signora Presidente, membri del Governo, colleghi, arriva finalmente in Assemblea un provvedimento di cui parliamo da molto tempo,

migliorato, con l'aiuto della Commissione e di tutti coloro che non politicizzano lo sport, perché lo sport è assolutamente autonomo, non è di destra, sinistra o centro e la maglia azzurra è la maglia di tutti. Per fortuna che è così, possibile, anche su argomenti di questo tipo, riuscire a fare errori che definire drammatici è poco. Faccio subito un esempio: quando si limita il mandato dei presidenti della federazione a due anni, non si pensa che quei presidenti rappresentano, esattamente come fanno gli atleti con la maglia azzurra, i dirigenti, il CONI, le federazioni, i ragazzi e tutto quello che c'è sotto tra cui i volontari - di cui parlerò dopo - e le famiglie, anche a livello internazionale? Uno diventava presidente della federazione,

gente che ci mette del suo. Questa era l'impostazione. Quando si votano i provvedimenti, ogni Gruppo decide come votare e naturalmente per noi farà la dichiarazione di voto il senatore Carraro, ma è giusto conoscere anche la storia dei provvedimenti. Questo è un provvedimento che è partito con errori madornali e solo il buonsenso e la disponibilità a sostenere un tema come quello dello sport, a cui non va dato colore politico, ha permesso finalmente che arrivasse in Aula migliorato.

i Gruppi. È ovvio che del CONI e dello sport bisogna occuparsi in un'autonomia totale. Ricordiamo un attimo cos'è lo sport e cos'è il CONI,

di cui il CONI giustamente si fa vanto, sono la punta dell'*iceberg*. Essi derivano dal lavoro svolto da questi volontari, dai tecnici, dagli educatori, perché spesso i maestri, i tecnici e gli allenatori sono educatori, insieme alle famiglie dei ragazzi, in queste società che stanno chiudendo.

Lo sport non si colora e non si può politicizzare, perché sarebbe un errore madornale, ma neanche si può farlo diventare burocrazia, perché lo sport è passione pura allo stato puro. È per questo che siamo riusciti a migliorare questo provvedimento: perché sappiamo di cosa parliamo. E non c'è bisogno di aver fatto sport a livello agonistico o aver fatto i dirigenti delle società sportive, basta guardare il mondo dello sport con l'occhio libero dall'ideologia,

colpiva le persone che fanno volontariato, dedicando se stesse alle società sportive. Immagino che i colleghi sappiano che i presidenti delle Federazioni vengono eletti dai presidenti delle società sportive,

rappresentato da persone che siedono anche in quest'Aula e che tanto hanno fatto per lo sport italiano e quindi per le famiglie e i ragazzi, perché non è che parliamo di famiglie e ragazzi quando ci fa comodo

sfaccettature. Io mi auguro che ci occuperemo di sport, come stiamo cercando di fare in 7a Commissione, in modo diverso. Perché allo sport va applicato il principio di sussidiarietà più puro, bello e semplice che esista,

È chiaro che il volontariato va aiutato, siamo tutti d'accordo. Ebbene, anche il mondo sportivo è volontariato all'ennesima potenza. Non fermiamoci a guardare la punta dell'*iceberg*, le medaglie e i risultati. Sotto quello c'è una grande montagna, c'è il sommerso, c'è quello che le famiglie vivono tutti i giorni. Quelle realtà sportive, quei dirigenti, quelle società sportive vanno aiutati, non ci si può fermare alle federazioni e non si poteva certo partire dalle federazioni in modo sbagliato perché siamo invasi dall'ideologia. Si è parlato di rottamazione dei volontari: ma credete che sia facile trovare un dirigente di società sportiva in qualsiasi città d'Italia e in qualsiasi piccolo Comune d'Italia?

le difficoltà che ci sono adesso nel Paese, le difficoltà economiche che hanno le famiglie? Non parlerò di questo, ovviamente, ma quando ne abbiamo parlato, abbiamo capito dove viviamo? Almeno quando parliamo di sport e volontariato cerchiamo di non chiudere gli occhi e di dirci come stanno davvero le

e cerchiamo di dare aiuto e di non parlare solo della punta finale dell'*iceberg,* ma anche di tutto quello che c'è sotto. che si occupa solo della punta dell'*iceberg* e ha detto che sotto c'è una grande montagna. In realtà, per occuparsi della grande montagna che sta sotto al mare noi dobbiamo partire, ovviamente, dal vertice. Lo sport è tema di grande rilevanza sociale ed economica e lo dimostrano i dati: 33 milioni di praticanti di cui 3,8 milioni nelle associazioni e società sportive e oltre 7,7 milioni negli enti di promozione sportiva, che davvero annoverano lavoro puramente volontario. Solo il CONI e le federazioni sportive contano 1.200 addetti, un indotto che coinvolge 35.000 imprese e 100.000 addetti con un valore aggiunto di 4,5 miliardi di euro e 14 miliardi di fatturato, ovvero circa il 5 per cento del PIL italiano. Un movimento di così grande vastità ha bisogno di avere una *governance* di grande efficacia, efficienza e soprattutto grande trasparenza. È in questa direzione che opera il testo di legge in esame, non solo intende garantire efficienza e credibilità alle istituzioni sportive del nostro Paese con il limite di mandati e deleghe, ma è un utile segnale di risposta alle istanze di rinnovamento della classe dirigente che sempre più spesso si levano dalla società civile. Lo scopo di questo testo è sottrarre le federazioni sportive nazionali a rischio di cristallizzazione nell'assetto gestionale. Per questo è fondamentale rivedere il sistema di rinnovo della dirigenza e dare garanzia dell'effettività del ricambio degli organi direttivi apicali. Questo serve ad una sana e corretta gestione di qualsiasi organismo pubblico, voglio ricordarlo, che si finanzi attraverso, appunto, soldi pubblici. Modificando il decreto-legge n. 242 del 1999 che disciplina il funzionamento del CONI e delle federazioni prevedendo, per queste ultime, un più chiaro e rigoroso limite alla durata complessiva dei mandati dei presidenti e dei consigli federali, si interrompono le interpretazioni e le prassi elusive dei limiti di legge, che pure c'erano. L'estensione del limite dei tre mandati per il Presidente ed i componenti di giunta nazionale del CONI e delle federazioni sportive, è esattamente in linea con la durata in carica del Presidente del CIO, il Comitato olimpico internazionale. Quindi, senatore Marin, in realtà noi, con questo testo, allineiamo del Presidente per otto anni rinnovabile una sotto volta per quattro. In questo modo l'ordinamento nazionale si adegua a quello internazionale. Altra cosa importante è quella di garantire un *turnover* finora bloccato all'interno delle federazioni sportive nazionali, dove - non nascondiamocelo - ci sono presidenti in carica dagli anni Novanta o dagli inizi del 2000, che, in alcuni casi eclatanti, sono giunti anche alla ribalta

la loro rielezione e legati alla creazione e alla gestione di associazioni e società sportive affiliate alle federazioni, in realtà fasulle, utilizzate come bacino di voti in occasione delle assemblee elettive federali, tramite il voto per delega.

che evita innanzitutto che le disposizioni possano essere poi annullate perché retroattive. Per evitare ricorsi sulla retroattività delle norme, si prevede che i limiti previsti dalla nuova normativa non si applichino a chi è in carica alla data di entrata in grazie a tutti Per quanto riguarda i limiti delle cinque deleghe, alcune federazioni dovranno rivedere anche gli statuti.

e rafforzato l'offerta formativa delle scuole, assumendo migliaia di insegnanti di educazione fisica per iniziare la pratica sportiva sin dalla scuola dell'infanzia e dalla scuola primaria. Si tratta di un provvedimento e di un'attenzione al mondo dello

Stiamo esaminando anche un affare assegnato che va ad esplorare tutti i punti sollevati durante questo dibattito parlamentare, dal lavoro sportivo, alla definizione sport dilettantistico e lo sport professionistico. Intendiamo davvero innovare con nuovi provvedimenti questo grande motore di crescita del nostro Paese. Caro senatore Marin, è vero che ci abbiamo messo tre anni per portare in Assemblea questo provvedimento; la invito allora a votare «sì» per la riforma costituzionale perché i provvedimenti di iniziativa parlamentare avranno senz'altro maggiori probabilità di vedere il traguardo in tempi certi. Ricordate, per favore, che è con quella riforma che noi possiamo valorizzare la democrazia parlamentare e non il contrario. Questo Paese, dunque, per risollevarsi e crescere ha bisogno di un maggiore tasso di innovazione e con questo provvedimento, cari colleghi, noi diamo nuovo impulso anche al mondo dello sport.

si influenzano a vicenda, stiamo discutendo in 7a Commissione, nell'ambito dell'affare assegnato sullo sport, di tutte le sfaccettature dello sport, per preparare Voglio ringraziare anch'io la Commissione, la capogruppo Puglisi, il presidente Marcucci e la sottosegretario Amici per il lavoro svolto insieme a tutti gli altri.

del ragionamento che ci ha accompagnato nel corso di un lavoro non semplice, abbastanza complesso e molto lungo. Anch'io, come la relatrice Idem,

il testo è molto circoscritto e riguarda un punto su cui si era rilevata una distonia nella norma transitoria, che era diventata l'elemento elusivo rispetto al decreto

abbastanza avanzato, che riguarda la disciplina dello sport di base, dove i temi sport, socialità, benessere e stili di vita attengono esattamente alla riflessione complessiva. Quando si affronta la tematica dello sport, a partire anche dai limiti di mandato, l'interesse e lo sguardo del Governo e della maggioranza che lo sostiene attengono a questa filosofia.

Guai a scindere gli impegni parlamentari, anche dentro argomenti circoscritti, dalla mancanza di visione. E questo - lo ricordava ora la senatrice Puglisi - è vero per quanto riguarda, ad esempio, alcune norme che abbiamo immesso nella buona scuola, con il recupero del valore dell'attività motoria e psichica dei giovanissimi, a partire dalle scuole elementari; abbiamo affrontato la questione dell'impiantistica, uno degli altri temi molto sentiti in questo Paese, facendo sì che l'impiantistica venga affidata anche alla gestione del CONI, con un'idea delle periferie che si lega al ragionamento del senatore Davico. Davico. Tutte queste questioni hanno un unico obiettivo: un Paese è competitivo quando si presenta nella scena e nella compagine internazionale con due condizioni, quando ha regole certe, applicabili e controllabili, e soprattutto una visione in cui non esistono solo gli aspetti economici o macroeconomici, ma anche

non italiani ma stranieri di aderire alle federazioni, a testimonianza che l'impegno dello sport parte proprio da questa capacità di inclusione dalla valorizzazione della socialità. *(Applausi

permettendo al mondo dello sport di avere un numero così alto di mandati e non ci sono dei limiti adeguati.

Signora Presidente, vorrei innanzitutto ricordare alla senatrice Puglisi che ci stiamo occupando di un disegno di legge e non della riforma costituzionale, infatti sul testo in esame cerchiamo di collaborare. Come ha detto

è evidente che cinque deleghe risulterebbero eccessive. Se ne potrebbero dare da due a cinque in base al numero degli associati.

non si vuole accettare questa minima tutela di onestà, di lealtà, di correttezza,

correttezza dello sport italiano? No. Non è possibile continuare su questa linea. Sin dal dibattito in Commissione abbiamo cercato In un primo momento si era accettato anche il limite di due mandati e il massimo di una delega. Ora le deleghe le abbiamo portate a cinque. Vogliamo almeno cautelarci dal punto di vista

Senatrice Petraglia,

non venga applicato alle associazioni di promozione sociale sportive o comunque alle altre associazioni sportive. Lo chiediamo perché diventa difficile districarsi per le associazioni sportive nella vastità delle vastità delle normative a cui devono sottostare. Nel corso degli anni, queste associazioni hanno dovuto adeguare i propri statuti a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 460 del 1997, così come dovranno fare della legge delega sul terzo settore, e di conseguenza aggiungere un ulteriore aggravio di adeguamento a una normativa che riguarda, oltre tutto, le federazioni del CONI. Questo ci sembra un eccessivo aggravio perché stiamo parlando - questo sì davvero - del volontariato sportivo di base diffuso sul territorio. Tra l'altro, vorrei ricordare che che in moltissimi statuti, proprio in virtù di quel piccolo margine di autonomia statutaria che questi riferimenti legislativi di cui parlavo

perché qualora uno statuto della federazione preveda un numero inferiore di mandati, è consentito di operare in tal senso.

inutile nascondersi che l'*iter* un po' travagliato di questo disegno di legge è stato incentrato sulla questione del numero dei mandati dei presidenti del CONI e delle federazioni sportive e territoriali. Su questo la difficile mediazione è stata finalmente risolta ricorrendo all'uso del buonsenso e anche della

di conciliare sensibilità diverse dal punto di vista culturale, dell'esperienza sportiva e del concetto che ognuno ha di sport, di pratica sportiva e del valore sportivo nella società, anche alla luce delle mutate esigenze di natura economica e sociale e dei contesti legislativi nazionali e internazionali.

dei fabbisogni delle federazioni piccole e grandi, di chi gode di buona salute nell'ambito delle organizzazioni delle organizzazioni sportive nazionali, e di chi invece (penso alle federazioni più piccole) mostra il fiato. Pertanto il numero di tre mandati ci sembra opportuno.

parere, mostrano anche un'altra faccia della medaglia (parlando di sport parliamo di medaglie), ovvero una maggiore responsabilità in capo al *management* dello sport, anche in vista di quella che appare essere la lunga stagione della candidatura di Roma, e quindi dell'Italia, ad ospitare le prossime Olimpiadi del 2024. il *management*, così rassicurato e tranquillizzato sul numero ampio di mandati, potrebbe lavorare affinché all'interno delle federazioni la pratica, la formazione, la preparazione, vengano eseguite con il massimo della serenità e dell'impegno. Questo significa anche raccogliere frutti, quanto più

Voglio inoltre raccomandare, a nome del Gruppo dei Conservatori e Riformisti, a seguito del nostro voto favorevole, la necessità che le federazioni, a cominciare dal CONI, si impegnino a formare sempre di più la classe dirigente dello sport in Italia. Tutte le discipline hanno bisogno di competenze vere, di competenze vere, che potrebbero offrire un'occasione di lavoro anche a quei laureati in discipline motorie motorie e in *management* e *governance* dello sport che nelle università italiane o straniere hanno acquisito il titolo.

nella professione a cui si candidano. In conseguenza di queste considerazioni e di questi ragionamenti, annuncio, a nome del

nel 2002. È un ente pubblico non economico, posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali,

cosa un po' simpatica che ho ricercato in questi giorni è che con la legge costituzionale n. 3 del 2001 si è avuta anche la riforma dell'articolo 117 della Costituzione con cui, per la prima volta, è stata inserita la parola «sport» all'interno del testo del nostro massimo atto normativo, anche indirettamente, che già l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'individuo non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali (tale è l'ordinamento sportivo ove si svolge la personalità

forte e pesante: la formazione del carattere, la prevenzione di alcune forme di malattia e la crescita dei ragazzi. Per quanto riguarda la questione legata

è ben attrezzata a svolgere un ruolo molto importante per i ragazzi. Forse bisognava mettere mano anche a quelle leggi che ancora oggi non riescono a supportare le attività

apprendere proprie di questi ragazzi, soprattutto in una certa area del nostro Paese. Abbiamo anche pensato che forse in una legge si poteva

tutti i presidenti delle associazioni sportive, a tutti i livelli, abbiano le stesse possibilità di essere noti sulla scena e di avere i riflettori dei *media* Ci sono tantissimi dirigenti che, a vario titolo, si occupano dei ragazzi e a volte è anche difficile trovare qualcuno che si impegni in modo serio e continuativo in quelle società minori che

avete cercato veramente di mettere in condizione chi deve approvare questa legge di essere convinto che sia una legge buona. Faccio solo due considerazioni: ho fatto qualche conto

Tra l'altro, per portare questo provvedimento in Assemblea si è impiegato circa tre anni. Vorrei chiudere semplicemente con una battuta alla senatrice Puglisi:

una legge che prevede lo spostamento da due a tre anni dei mandati del Presidente del CONI (e qualcuno in quest'Aula ha sostenuto anche che il testo originale non era proprio il massimo della vita e ha subito parecchie modifiche per essere migliorato), dico semplicemente che, senza il bisogno di eliminare una delle due Camere, si sarebbe un disegno di legge più serio all'inizio e forse magari, in un paio di mesi, si sarebbe risolto il problema. Con queste considerazioni

MPL))*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come dicevo in discussione generale, è imbarazzante oggi dover dedicare questo voto solo al limite dei mandati. Non sto sminuendo il valore di questo testo di legge, che in fondo è una maniera di occuparci dello sport in quest'Aula. Purtroppo, siamo di fronte a un tentativo di innovare una questione ormai degenerata,

è proprio l'esempio che documenta come oggi il CONI non sia più tutto lo sport e come lo sport non sia solo il CONI. Almeno questo avviene nella realtà, tutti i giorni, nelle grandi aree metropolitane e nei piccoli paesi. Ci stiamo oggi occupando di burocrazia e *governance* o di sport? dobbiamo ricordare che è sport, attività sportiva, quella sulle spalle delle nostre famiglie che, quando desiderano inserire un'attività sportiva nell'educazione dei loro figli, devono rivolgersi a quelle migliaia di volontari, grazie a tutti

Facciamocene carico, e non solo attraverso gli investimenti cui la collega Puglisi opportunamente faceva riferimento. Resta il problema dello sport sociale, dello sport di base,

oggi annuncio il mio voto di astensione su questo provvedimento, in polemica con la leggerezza con cui ci si occupa del CONI e dei massimi vertici nazionali del nostro sport. Resto in attesa di risposte (e vi ho già accennato prima) su questa auspicabile riorganizzazione delle nostre politiche sportive, socio sportive, socio culturali sportive.

Signor Presidente, abbiamo ascoltato, negli interventi in discussione generale, parole molto interessanti sull'alto valore dello sport. Tutti noi riconosciamo il particolare valore dello

d'accordo. Lo sport è una parte importante del *welfare* e della coesione sociale, perché abbatte barriere discriminatorie e favorisce l'integrazione. Pensiamo alla facilità con cui lo sport favorisce l'inserimento sociale come lo sport aiuti nell'accoglienza, nel confronto con gli altri, nel costruire la dimensione collettiva. Lo sport aiuta nella lotta contro l'illegalità e contro le mafie, perché lo sport è regole e gioco e i due aspetti sono molto collegati tra di loro. Penso al ruolo che lo sport ha nella crescita dei ragazzi e all'importanza di dover investire, sin dalla prima infanzia, a partire dalla scuola, nello sport. In questi anni, però, abbiamo sentito parlare poco di tutto questo da parte dei Governi perché poco si sono dedicati allo sport, e soprattutto poco allo sport di base, a quello che dovrebbe essere garantito a tutti. L'attenzione spesso è stata concentrata sui grandi eventi e sulla costruzione di grandi impianti. Sono state investite ingenti risorse per la costruzione di impianti sportivi, spesso inutilizzati e non completati, creando dei veri e propri mostri di cemento nelle città, senza pianificazione urbanistica, e che spesso, troppo, hanno prodotto corruzione negli appalti. Storie recenti. Abbiamo visto costruire impianti nuovi in città dove non sarebbero necessari e niente invece è stato investito per la costruzione di impianti sportivi, anche piccoli purché sufficienti e utili, nei piccoli centri, al Sud, nelle periferie, dove la promozione della pratica sportiva avrebbe un valore immenso di inserimento e uguaglianza sociale. Ecco, noi oggi avremmo voluto che l'Aula del Senato, che si riunisce per la prima volta per parlare di sport, avesse avuto modo di parlare di questo. Invece ciò non avviene perché, ovviamente, ci saremmo dovuti trovare dinanzi ad un atto di iniziativa parlamentare o del Governo, ma questo Governo, vorrei ricordarlo, non ha un Ministero dello sport. Dopo la parentesi della delega Delrio, noi ancora oggi non sappiamo ufficialmente chi segue lo sport, senza nulla togliere alla Sottosegretaria presente, che ovviamente il primo atto che oggi discutiamo riguarda un disegno di legge sui mandati del CONI. Ci è stato detto che bisogna occuparsi della *governance* prima della marea, delle acque e delle montagne. Insomma, è chiaro, ci sembra evidente e lo abbiamo visto anche nella discussione in Commissione, che c'è un vero e proprio tentativo di trasferire le funzioni del Ministero dello sport al CONI. Questo, ovviamente, è molto grave. Oltre tutto, stiamo parlando di un ente che gestisce milioni di fondi. La Commissione, in questo periodo, è impegnata in una discussione su un affare assegnato sullo sport, quindi stiamo ascoltando il variegato Per questo sarebbe stato utile parlare di molto altro e invece oggi ci troviamo, dopo un lavoro in Commissione - qualcuno lo ha ricordato - durato circa tre anni, di lunga mediazione e di lunga discussione di cui confesso non abbiamo nemmeno ben compreso il senso,

ci siamo ritrovati qualche giorno fa, con questo disegno di legge iscritto all'ordine del giorno dell'Aula da mesi,

Non è un caso che il cambio dei tre mandati, è stato già detto da chi mi ha preceduto, sia sicuramente un modo per allineare la discussione con quello che accadrà nel 2024 se Roma dovesse se Roma dovesse essere il luogo dove si faranno le Olimpiadi. Ovviamente tutto questo impatta con quanto accaduto nelle ultime settimane con le elezioni amministrative. Non siamo così stupidi da non capire ciò che grazie a tutti di riformare i grandi enti che gestiscono - ripeto - importanti e sostanziali risorse pubbliche. Per questo motivo, dichiaro il voto contrario di Sinistra italiana.

l'*iter* a cui è andato incontro è stato invece indubbiamente lungo, iniziato in 7a Commissione a gennaio 2014, conclusosi a settembre 2015, per andare incontro poi ad una lunga pausa in Conferenza di capigruppo, prima dell'approdo in Non c'è dubbio che l'*iter* lungo e alquanto travagliato di questo provvedimento è sintomatico di quanto diversificate siano le posizioni su questi temi. Devo dare atto alla relatrice di essere riuscita, nonostante le molte perplessità ed in alcuni casi anche resistenze, a portare all'approvazione questo disegno di legge dopo un paziente lavoro di mediazione e di conciliazione di aspettative, posizioni e interessi diversi. Porre un limite massimo al numero di mandati ai vertici del CONI e delle varie federazioni sportive non risponde ad una logica di ricambio fine a se stessa, bensì all'esigenza di portare idee innovative e nuove energie quanto mai necessarie nella gestione degli organismi sportivi. Questo fattore si ritiene essere particolarmente importante per gli enti di promozione sportiva, per gli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, dove molto spesso l'attività dei dirigenti è svolta essenzialmente in forma del tutto volontaria e dove il permanere troppo a lungo delle figure dirigenziali può essere limitante della necessità di ampliare il coinvolgimento nella gestione delle attività. È un principio che sembra cozzare con la necessità di grande esperienza, soprattutto a livello internazionale, dove contano molto i rapporti, la credibilità, le collaborazioni, le alleanze per consentire ricadute positive a livello interno. Rapporti, collaborazione, credibilità si acquisiscono però con il tempo, con il consolidamento delle relazioni stesse; per questo non applicare la retroattività, come previsto nel provvedimento originario, consente di assorbire in maniera graduale, quindi non traumatica, la nuova previsione del limite al numero di mandati. E questo assume un significato particolarmente importante essendo in corso le candidature di Cortina per i Mondiali di sci del 2021 e di Roma per le Olimpiadi del 2024. Il secondo tema che affronta questo disegno di legge è quello relativo al numero di deleghe che si possono esercitare. Effettivamente il numero di 40 previsto dal CONI anche per le altre federazioni, è elevato, probabilmente eccessivo. Il limite proposto di 5 chiama tutti i responsabili delle associazioni ad una maggiore partecipazione, più diretta e responsabile, senza creare problemi di gestione delle assemblee direttive, che è stata una perplessità sollevata dalle attuali dirigenze. Dire che lo sport in Italia è un fenomeno sociale con grande rilevanza anche da un punto di vista economico non è azzardato; è la semplice fotografia della situazione questo provvedimento si inserisce in un momento in cui, senza sminuire l'importanza che lo sport ha avuto anche negli anni scorsi, si sta assistendo (richiamo dati Istat, quindi dati ufficiali), dopo qualche anno di flessione, ad una ripresa della pratica sportiva, soprattutto della pratica di base, quella a livello scolastico e giovanile, e anche da parte della fascia di persone della terza età. Secondo il recente studio Istat, l'aumento si registra in tutte le classi di età, ma con una crescita più decisa fra i bambini di sei-dieci anni (dove la quota passa da 59,5 per cento a 65,3 per cento) e fra le persone che risiedono in Comuni centro dell'area metropolitana.

le quote femminili scendono invece a 19,5 per cento e a 7,7 per cento. Solo fra i piccolissimi (tre, cinque anni) vi è un'incidenza maggiore di bambine che fanno sport, aspetto che fa ben sperare per il futuro. La pratica sportiva dei genitori, inoltre, influenza positivamente la pratica sportiva dei figli. Sono dati che devono essere analizzati con attenzione sia a livello politico, sia a livello di amministrazioni locali, sia da parte delle federazioni e delle associazioni sportive per programmare, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità nuovi scenari per lo sport italiano. Dico questo riferendomi anche all'indagine che sta effettuando la 7a Commissione - citata prima dalla relatrice Idem - sullo stato dello sport in Italia, che presumo si concluderà prima dell'estate, dopo una lunga serie di audizioni che hanno consentito di sviscerare a 360 gradi tutte le problematiche dello sport, con un documento che fornirà indicazioni e prospettive per le future politiche sportive in Italia. Il voto di Area Popolare a questo disegno di legge sarà favorevole.

ed è praticato da 13 milioni di italiani. Questo disegno di legge poteva avere un valore fortemente simbolico, perché la sua *ratio* originaria convergeva con una delle proposte cardine del Movimento 5 Stelle, cioè il limite inderogabile dei due mandati per i più importanti incarichi pubblici, dal parlamentare ai gradi apicali di enti o società pubbliche. si intendeva dare un limite temporale anche all'incarico del Presidente del CONI, dei componenti degli organi direttivi apicali e dei presidenti e vertici delle federazioni sportive, oltre che delle discipline sportive associate. In sede di 7a Commissione abbiamo lavorato molto per cercare di mantenere questa iniziale impostazione, che avrebbe sicuramente rappresentato un forte cambiamento a tutti i livelli nella gestione degli organismi di autogoverno dello sport, nonché contribuito da subito a sottrarre il CONI e le federazioni sportive nazionali dal controllo di quelle classi dirigenti che per lunghi periodi hanno governato lo sport italiano, cristallizzandone la gestione con con logiche di spartizione direttamente associabili ai partiti tradizionali. Tuttavia, siamo riusciti solo parzialmente a raggiungere l'obiettivo, perché dopo l'approvazione in 7a Commissione di un emendamento a mia prima firma, con cui si stabiliva, si stabiliva, in modo più chiaro rispetto al testo originario, il limite dei due mandati, nonché il divieto, per l'elezione dei presidenti e dei membri degli organi direttivi

di svolgere ulteriori due mandati, se eletti. Già questa norma era stata prevista dalla relatrice Idem, con l'indicibile ma chiaro obiettivo di ritardare quel ricambio generazionale di cui il nostro Paese invece ha bisogno, anche nello sport, nonché di rinsaldare quelle rendite di posizione e quei meccanismi che ormai da decenni assicurano una gestione elitaria dello sport. Per questo motivo avevo proposto in Assemblea un emendamento che stabiliva l'inapplicabilità della norma transitoria per coloro che ricoprono, da almeno dieci anni, sia a livello nazionale che territoriale, incarichi apicali nell'ambito del CONI e delle federazioni sportive, in modo da creare un vero è proprio «anno zero» per i vertici dello sport e favorire, appunto, quella ventata di aria nuova che solo un vero ricambio generazionale può garantire. Cari colleghi del Partito Democratico, in questi tre anni di governo avete predicato bene e razzolato male, avete parlato da rottamatori e agito da restauratori. Infatti, se analizziamo l'azione politica di questo Governo, non è difficile comprendere come il *premier* Renzi, appena insediatosi a Palazzo Chigi, abbia rottamato le sue idee invece dei poteri forti, con i quali continua a fare accordi. Un'ulteriore conferma in tal senso è pervenuta con il disegno di legge quando proprio ieri la relatrice Idem, con la quale inizialmente si erano create le condizioni per lavorare proficuamente, è stata costretta ad abbandonare i buoni propositi di collaborazione e a chinare il capo di fronte alle logiche ricattatorie che governano il Partito Democratico, presentando alcuni emendamenti che stravolgono totalmente il disegno di legge inizialmente previsto, inserendo la possibilità per il Presidente del CONI e i componenti della giunta nazionale di svolgere tre mandati e non più due, nonché la possibilità all'interno delle assemblee elettive di poter esercitare fino a cinque deleghe e non più una, come invece avevamo giustamente ottenuto in Commissione. Sono scelte, queste, che dimostrano la volontà del Governo e del Partito Democratico di non garantire la normale alternanza delle cariche presidenziali e dirigenziali nel mondo dello sport, bensì di cristallizzarle, come se lo sport fosse una questione privata, quasi personale, sulla quale i partiti sono interessati esclusivamente a esercitare, ai fini dei consenso, la loro influenza e il loro potere, anche con l'esclusiva presenza del CONI all'interno delle scuole. Dopo questi accordi, ben evidenziati dal ritiro di tutti gli emendamenti del senatore Carraro, sono state rifiutate le modifiche proposte alla collega Idem con subemendamenti a nostra firma che reintroducevano il limite dei due mandati e che legavano il quantitativo di deleghe da esercitare al numero degli associati delle singole federazioni nazionali e delle discipline sportive associate.

di esprimere al massimo due preferenze per gli organismi dirigenti del CONI e delle federazioni nazionali, indispensabile per garantire maggiore trasparenza e democrazia nel mondo dello sport, ma che certamente andava a cozzare con quella pericolosa visione che vede

che permette alle parti di alimentarsi reciprocamente. Considerate, ad esempio, l'eventuale assegnazione alla città di Roma dei giochi olimpici del 2024. L'attuale presidente del CONI Giovanni Malagò ha annunciato, nel caso in cui Roma ottenesse i giochi, di volere la costruzione del nuovo villaggio olimpico a Tor Vergata: aree verdi che si vorrebbero interamente edificate, si parla addirittura di 15.000 appartamenti *ex novo*, per la gioia degli influenti palazzinari romani. Ma Roma adesso è governata dal Movimento 5 Stelle e se anche volevate fare il piano casa a Roma, il tempo delle vacche grasse è finito, è finito! Abbiamo Roma e 12 municipi! Se si ha, quindi, contezza di questo scenario, dei molteplici interessi che gravitano attorno allo sport e, infine, del fatto che il provvedimento in esame, con il solito colpo di mano della maggioranza, si è trasformato nell'ennesimo *bluff* dell'era renziana (ormai agli sgoccioli), si comprendono bene i motivi che ci portano a continuare la nostra battaglia di trasparenza e democrazia alla Camera e a votare adesso convintamente no. Signora Presidente, signora Sottosegretario,

nel corso di questi tre anni, che sono stati ricordati. Vorrei anche ringraziarli per il fatto che stanno cercando di approfondire con grande serietà

Per esempio, c'è un problema che riguarda le donne: da una parte le donne partecipano alle Olimpiadi per il 47 per cento - la partecipazione femminile è pertanto consistente

il suo ciclo; adesso però è vero che il CONI prende 400 milioni dallo Stato con la legge di stabilità, ma è altrettanto vero che dalle sole scommesse sportive lo Stato ricava Pertanto, ancora oggi, se consideriamo quanto lo Stato investe a livello centrale e periferico e quanto lo sport produce,

delle associazioni non riconosciute dell'attività paralimpica sono volontari che, solo in taluni casi, prendono rimborsi spese.

perché la crisi economica fa sì che la gente abbia meno tempo a disposizione e meno denaro per anticipare le spese dei giovani che devono partire. Non voglio dilungarmi per spiegare un meccanismo che conoscete. Sul numero dei mandati

"Francois Carrare", l'autore di questa riforma, ha spiegato alla Commissione cultura del Consiglio d'Europa, di cui alcuni senatori fanno parte,

collaborano con le società sportive, con qualche scuola, e ci si arrangia anche a coprire vuoti che in realtà esistono. Queste società sportive spesso sono bloccate, paralizzate nella loro attività per pastoie burocratiche e formalismi fiscali che non portano soldi allo Stato ma creano problemi notevoli ai loro dirigenti. Oggi approviamo un provvedimento serio. Non fermiamoci qui. Cerchiamo soprattutto di aiutare le società sportive di base.

Abbiamo l'opportunità di parlare nuovamente di sport. Dico nuovamente perché, grazie al Governo, grazie a tutti noi, recentemente abbiamo parlato di interventi sulle infrastrutture sportive; abbiamo parlato di inclusione - lo ricordo - in particolare rispetto ai minori, attraverso provvedimenti di buonsenso. Stiamo lavorando sulle scuole. Ricordo che la riforma della scuola

Quindi, si arriva a fare processi normativi, anche complessi, che hanno avuto bisogno di approfondimenti, di comprensione. Però - lo dico come rappresentante del Partito Democratico - io mi prendo il merito. I miei colleghi hanno il merito, nello specifico, di aver sollevato la questione

per la formazione e l'educazione dei nostri giovani, con la sua prepotente funzione sociale, anche di inclusione.

*(M5S)*. Signor Presidente, era il 1979 quando il Comune di Somma Vesuviana assegnò alla Soficoop SpA

liquidazione) la realizzazione di abitazioni nell'ambito di un bando regionale per l'edilizia agevolata. Venne assegnato alla Soficoop, oltre alla costruzione e alla vendita degli immobili, anche il compito di occuparsi degli espropri dei terreni e dei relativi indennizzi ai proprietari. Al Comune restava la responsabilità di vigilare sul corretto svolgimento di tutti questi processi. Sul lato degli immobili, gli assegnatari versarono alla Soficoop una caparra di 80 milioni delle vecchie lire; i restanti 60 sarebbero stati erogati attraverso un mutuo da stipulare con il Banco di Napoli. terreni, però, ai proprietari non venne mai corrisposto dalla Soficoop alcun indennizzo. Quali sono state le conseguenze? Non è mai stato possibile per gli assegnatari chiedere i mutui (sebbene avessero versato alla Soficoop) e stipulare quindi i contratti definitivi, perché la Soficoop, non avendo provveduto agli espropri (mentre il Comune dormiva),

che avevano fatto causa; l'operazione è costata tre milioni di euro alle casse del Comune (e dei contribuenti sommersi, ovviamente). La Soficoop è attualmente in liquidazione e sugli appartamenti è partita una procedura di recupero crediti

in un'iniziativa che doveva essere sulla carta un processo agevolato e che si è trasformata, per una somma di inefficienze

A fine giugno sono previste le prime aste e i successivi sgomberi: un incubo senza fine. Abbiamo presentato un'interrogazione ai Ministeri

Signor Presidente, ieri, nel mio intervento di fine seduta, ho parlato della vicenda della bimba vegana di Genova. Ebbene, nel mio intervento di ieri ho avuto la possibilità di citare il mio discorso discorso telefonico con il direttore sanitario dell'ospedale Gaslini di Genova, che mi aveva riferito che la bambina, durante la fase dello svezzamento, aveva anche mangiato parmigiano. Questo toglie qualsiasi dubbio

Nel mio intervento di ieri ho citato anche un caso precedente, del 15 ottobre (ieri ho parlato erroneamente di Treviso, ma in realtà si trattava del caso di Belluno). Anche in quel caso, il 15 ottobre contattai il direttore medico della direzione sanitaria dell'ospedale di Belluno, che chiarì in maniera inequivocabile la questione. Mentre i giornali continuavano a scrivere «Bambino vegan in ospedale: nuovo caso a Belluno», in realtà il direttore medico mi chiarì che

pubblicitaria del Ministero delle politiche agricole "Ora del latte". È infatti intervenuto l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria ed ha fatto cambiare le pagine del sito pagato con soldi pubblici. Inoltre, l'organismo di regolamentazione pubblicitaria ha scritto, sulla base della documentata denuncia scientifica, l'apporto proteico e di nutrienti fornito dal latte di mucca può essere sostituito senza inconvenienti da altri cibi non di origine animale. Credo pertanto che sia ora di farla finita con questo attacco a chi ha scelto consapevolmente di seguire un'alimentazione completamente vegetale che, come ripeto

Signor Presidente, apprendiamo dagli organi di stampa oggi che una sentenza del TAR Lazio, a seguito di un ricorso presentato da alcune associazioni teatrali, tra cui il Teatro Elfo Puccini di Milano e il Teatro Regio di Parma, ha abrogato il decreto ministeriale dell'agosto 2014 che interveniva sui meccanismi di ripartizione dei finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo relativamente allo spettacolo dal vivo. un provvedimento che era stato scritto da una manina nota all'interno del Ministero e anche al mondo dello spettacolo dal vivo, ossia quella dell'ex direttore generale Salvatore Nastasi. Alla notizia dell'emanazione di questo decreto ministeriale, il mondo dello spettacolo dal vivo era insorto, perché all'interno del provvedimento si introduceva come meccanismo di funzionamento un algoritmo, che oggettivamente avrebbe dovuto stabilire quali associazioni sarebbero state beneficiarie dei finanziamenti, eliminando quindi qualunque criterio di soggettività basato sulla valutazione delle commissioni.

Ebbene, noi abbiamo presentato un'interrogazione ed abbiamo fatto presente al ministro Franceschini che questo decreto ministeriale era negativo perché avrebbe sancito la morte di tante realtà culturali. Addirittura abbiamo richiamato l'attenzione del ministro Franceschini Franceschini sulle dimissioni di Silvia Colasanti dalla commissione musica, presentate per protestare non solo per il funzionamento della commissione, ma anche contro i meccanismi introdotti dal suddetto decreto. Il ministro Franceschini però non ci ha voluto ascoltare, come al solito, e non ha voluta neanche ascoltare l'appello degli artisti, che hanno raccolto 3.500 firme. Anzi, ricordo benissimo che in una delle ultime audizioni in cui il Ministro è stato richiamato su questi fatti, ha vi piaccia o non vi piaccia, così è. Il Movimento 5 Stelle si appresta a presentare un'interrogazione, perché chiaramente questa sentenza di fatto abroga quel decreto ministeriale, probabilmente bloccherà l'erogazione di questi finanziamenti e paralizzerà un sistema. Abbiamo letto che tutto ciò è al vaglio della direzione generale dello spettacolo dal vivo. Presenteremo un'interrogazione per chiedere al Ministro delle attività culturali che cosa intenda fare e se questa volta intenda consentire un passaggio parlamentare come si deve, coinvolgendo le Commissioni competenti. Speriamo di non ricevere una risposta risposta desolante e che poco si adegua alla figura di un Ministro, che è quella appunto: vi piaccia o non vi piaccia, così è. Ne prenda atto, ministro Franceschini.